La seduta è aperta

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

il Governo intende doverosamente informare il Parlamento circa i recenti sviluppi relativi a un *asset* strategico di rilievo nazionale e internazionale, perché siamo in un momento decisivo che richiama tutti al massimo senso di responsabilità. Questa sera la delegazione di Governo farà altrettanto nell'incontro con le rappresentanze sindacali, con cui ci siamo spesso confrontati in questo anno, sin dall'inizio della legislatura; rappresentanze sindacali che ben conoscono lo stato della situazione e l'urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi dieci anni. Gli impianti siderurgici dell'ex Ilva di Taranto, con i suoi stabilimenti anche in Liguria, hanno segnato in oltre sessant'anni la storia - potremmo dire davvero - l'epopea della siderurgia italiana, con il lavoro e il sacrificio di intere generazioni e, purtroppo, anche con le conseguenze che ben conoscono gli abitanti del quartiere Tamburi, a cui vanno il nostro pensiero e il nostro impegno affinché si possa davvero completare il processo di riconversione ambientale dello stabilimento. L'ex Ilva, primo impianto di acciaio primario in Europa, ha consentito al nostro Paese di realizzare un sistema industriale che ha portato sviluppo e benessere e ci consegna al secondo posto, dopo la Germania, nell'Unione europea. L'Italia delle autostrade e delle auto, l'Italia della nautica e della cantieristica, l'Italia degli elettrodomestici, della meccanica, delle ferrovie, delle infrastrutture e delle costruzioni esiste in quanto può contare sulla sua importante e significativa filiera siderurgica. Noi ci crediamo e ci impegniamo a ricostruirla competitiva sulla tecnologia *green* su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa. Tutti voi sapete che l'impianto è in una situazione di grave crisi. Per quanto riguarda la produzione si attesterà - non abbiamo ancora i dati complessivi - a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l'obiettivo minimo che nel 2023 avrebbe dovuto essere di 4 milioni, per poi quest'anno risalire a 5 milioni. Nulla di quello che era stato programmato e concordato è stato realizzato. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale. In questi anni la produzione si è progressivamente ridotta, in spregio agli accordi sottoscritti. Persino negli anni in cui la produzione di acciaio era altamente profittevole in Europa, come nel 2019, la produzione è stata mantenuta bassa lasciando campo libero ad altri attori stranieri che hanno aumentato invece la loro quota di mercato in Italia. Noi intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio e delineando un piano siderurgico nazionale che sia costruito su quattro poli complementari, attraverso un progressivo percorso di rinnovamento, modernizzazione e specializzazione degli impianti esistenti. Mi riferisco *in primis* appunto a Taranto, che dovrà riaffermare il ruolo di campione industriale con una filiera produttiva con l'intero ciclo dal minerale al prodotto finito. Mi riferisco a Terni, dove lavoriamo sul solco di quanto fatto dal mio predecessore Giorgetti, per il rafforzamento della produzione di acciaio speciale con un contratto di programma che dovrebbe essere definito entro febbraio. Mi riferisco a Piombino, con l'enorme potenzialità, in particolare sulle rotaie, che fin qui ha sottoperformato e che ora registra l'interesse, oltre che del soggetto presente, di potenziali nuovi investitori stranieri con i quali ci apprestiamo a sottoscrivere un *memorandum* d'intesa per il riavvio della produzione di acciaio. Da ultimo, ma primo per importanza di produzione, cito il supporto alle acciaierie, soprattutto nel Nord, che stanno portando avanti con successo una svolta *green* senza precedenti, modello di efficienza sostenibile in Europa, e dobbiamo dare atto ai nostri imprenditori dei grandi sforzi fatti. Si tratta, quindi, di un piano articolato, che ovviamente dovrà tener conto anche del contesto europeo e delle misure competitive messe in campo dagli altri attori globali

fra acciaio verde e acciaio inquinante, è un elemento di riequilibrio necessario ma non ancora sufficiente. Il CBAM, infatti, mira a porre oneri economici sui produttori esteri che lavorano in Paesi a minore onerosità di utilizzo dell'anidride carbonica, ma da solo non basta a ridare competitività alle imprese europee, che infatti hanno ridotto i loro programmi di investimento e alcuni, come appunto Mittal (il più grande attore globale), ci hanno detto con chiarezza che a queste condizioni investiranno negli Stati Uniti e non certo in Europa. Dobbiamo quindi intervenire anche in quella sede, a Bruxelles, e lo faremo, per garantire migliori condizioni di produzione e quindi di investimento in Europa, anche per salvaguardare l'autonomia strategica del nostro continente e quindi la sua competitività globale. Avevo il dovere di chiarire il contesto non solo perché dobbiamo definire finalmente una politica industriale duratura nel tempo, al di là delle legislature, ma anche perché dobbiamo dire per quale motivo siamo arrivati a questo punto e cosa abbiamo fatto in questo anno di Governo per riprendere in mano la situazione di quello che è un bene di tutti gli italiani e certamente dei lavoratori metalmeccanici e delle loro famiglie che vi hanno dedicato la loro vita e che non vogliamo assolutamente deludere. Il loro lavoro va onorato con il nostro impegno. Noi non siamo condizionabili, come non lo sono loro, perché sappiamo cos'è la fatica del lavoro e perché ricordiamo che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Ricordo quindi a voi tutti e a me stesso come si è giunti a questo non per recriminare, ma per rimediare; non per accusare, ma per superare, spero insieme. Nel gennaio 2016 era in carica il Governo del collega senatore Renzi; gli allora commissari dell'amministrazione straordinaria ritennero di bandire una gara per la vendita dell'*asset*, centrata su alcuni elementi di rilievo ambientale, industriale e ovviamente anche economico.

La multinazionale indiana ArcelorMittal, primo attore globale, vinse la gara pubblica per assumere in affitto la gestione delle acciaierie, in attesa dell'acquisizione, pur in presenza di un'altra cordata pubblico-privata cui partecipava perfino Cassa depositi e prestiti, la mano dello Stato.

nell'anno in cui conveniva produrre gli acciai in Italia e in Europa, un anno grandemente profittevole per le acciaierie, sempre con il Governo Conte I - Ministro dello viene tolto lo scudo penale e ArcelorMittal rende nota di conseguenza la propria intenzione di sciogliersi dall'accordo. Ricordo che in quella circostanza numerose voci si levarono dall'opposizione di allora anche in quest'Aula del Senato e personalmente fui una di quelle. Mi alzai in quest'Aula per affermare, a nome del partito cui appartengo, che la rimozione dello scudo penale in un contesto come quello di Taranto avrebbe giustificato il disimpegno della multinazionale indiana, che peraltro, secondo i secondo i più, aveva fatto quell'investimento non per rilanciare l'impianto, ma per evitare che potesse rappresentare una concorrenza di mercato dall'Italia in Europa. Quella decisione sulla rimozione dello scudo penale pose ArcelorMittal in una posizione di forza nei confronti del Governo di allora. Di fronte alla minaccia di abbandonare il sito e in assenza di alternative, nel marzo 2020 il Governo Conte II - Ministro era allora il collega senatore Patuanelli - avvia una nuova trattativa con gli investitori franco-indiani, da cui nascerà Acciaierie d'Italia, con l'ingresso di Invitalia al 38 per cento e con la sigla di patti parasociali fortemente sbilanciati a favore del soggetto privato; patti che definire leonini è un eufemismo. Nessuno che abbia cura dell'interesse nazionale avrebbe mai acconsentito a quel tipo di accordo; nessuno che abbia conoscenze delle dinamiche industriali avrebbe accettato mai quelle condizioni. La *governance* era di fatto rimasta nelle mani del socio privato, che nel frattempo però deconsolidava l'*asset*, a dimostrazione del proprio disimpegno, richiamando anche i propri tecnici e non immettendo più alcuna risorsa nell'azienda. In particolare, all'amministratore delegato designato da Mittal è stato riconosciuto il voto decisivo su ben sette materie di straordinaria importanza per la vita dell'acciaieria; al presidente designato da Invitalia, invece, il voto decisivo su una sola materia. Anche nell'ipotesi prevista in quella intesa inizialmente per il maggio 2022 e poi spostata a maggio 2024, cioè al maggio di quest'anno, di una salita in maggioranza del socio pubblico al verificarsi di alcune condizioni, Invitalia comunque non avrebbe potuto designare un amministratore di proprio fiducia. Ripeto: anche se fosse diventata maggioranza, Invitalia non avrebbe comunque potuto esprimere un amministratore di propria fiducia, come ha recentemente dichiarato proprio il socio privato, rivendicando ancora l'altro ieri, in una dichiarazione ufficiale alla stampa, condizioni di privilegio garantite da quei patti.

Unica possibilità concessa era quella di cedere non più del 9 per cento, quindi scendendo dal 60 al 51, a un socio finanziario, non industriale, non operativo sull'acciaio e comunque con diritto di prelazione in capo a Mittal. In questa situazione, compromessa da un accordo sottoscritto in condizioni di minorità, ci siamo mossi sin dall'inizio nel cercare di recuperare allo Stato margini di azione e nel contempo per tentare di invertire la rotta del declino produttivo e ogni intervento in questo anno, sin dal decreto sull'ex Ilva realizzato alla fine del 2022, è stato in questa direzione. Con il decreto Ilva del dicembre 2022 abbiamo introdotto la non punibilità in caso di *asset* dichiarati di interesse strategico nazionale per azioni che discendono dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento, dirette a tutelare i beni giuridici protetti. Abbiamo sostenuto il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia con 680 milioni di euro convertibili in azioni in qualunque

Abbiamo messo a disposizione di Invitalia un ulteriore miliardo di euro per sostenere eventuali esigenze finanziarie aggiuntive della società che si rendessero necessarie per raggiungere gli obiettivi produttivi per il 2023 indicati concordemente in 4 milioni di tonnellate di acciaio, come deriva dal concordato nel *term sheet*, che nel frattempo è stato definito concomitante al decreto-legge. Abbiamo inoltre previsto la possibilità che il socio pubblico possa intervenire, ove vi siano le condizioni di insolvenza, attraverso le procedure di amministrazione straordinaria, ove queste non le attivasse doverosamente il rappresentante legale. È una sorta di catenaccio, quella norma, per tutelare comunque il bene pubblico. Con la finalizzazione degli accordi di gennaio 2023 tra i soci, abbiamo ridefinito parzialmente - e ripeto parzialmente - i precedenti accordi, realizzando migliori condizioni di *governance* e prevedendo il possibile ingresso di un altro attore industriale, anche in *partnership* (cosa in precedenza espressamente esclusa). Abbiamo inoltre fatto in modo che, entro la fine di febbraio dell'anno appena trascorso (2023), fossero rese disponibili le quote dei certificati ETS gratuite spettanti alla società, con significativi benefici finanziari stimabili nell'ordine di 250 milioni di euro. Abbiamo sbloccato l'istruttoria dei contratti di sviluppo, creando le condizioni per gli ulteriori investimenti di decarbonizzazione, oltre a quelli relativi agli investimenti industriali (*revamping* di altoforno 5, il più grande altoforno d'Europa, interventi su altoforno 4, altri interventi) e alla realizzazione del forno elettrico. Abbiamo da ultimo introdotto con il decreto *asset* - i colleghi senatori lo ricorderanno - la possibilità di cessione degli impianti pur in vigenza di sequestro, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui l'ultimo grado di giudizio dovesse confermare la confisca degli impianti. Questa norma è strategica per chiunque gestirà l'impianto La possibilità di acquisire gli impianti e la conseguente patrimonializzazione possono portare a una pronta bancabilità e quindi alla liquidità per l'azienda indispensabile per assicurare le manutenzioni e gli investimenti, nonché per il riavvio delle produzioni. Come si vede, lo sforzo che le istituzioni (il Governo e il Parlamento) hanno condotto in questi mesi è stato orientato a creare le condizioni per un maggiore impegno degli azionisti, delineando anche a più riprese quali sono le priorità per l'ex Ilva dal punto di vista della produzione e dell'occupazione. Abbiamo a più riprese chiarito al socio privato come sia necessario un impegno congiunto sui fabbisogni immediati, sulla ricapitalizzazione, sull'acquisto degli *asset* e sugli investimenti produttivi e ambientali. Occorrono interventi straordinari di *revamping* di alcuni altiforni, il rifacimento degli impianti che servono per trasformare in energie i gas di altoforno, l'installazione di un forno elettrico con l'utilizzo del preridotto (DRI) a minor impatto ambientale, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di trasformazione, laminatoi, tubificio e centri di lavorazione dislocati a Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi e altri centri minori; il completamento della messa in sicurezza e della bonifica, laddove necessaria, delle aree, anche in funzione di possibili alternativi utilizzi a vantaggio della comunità locale. Come è noto, il Governo ha incontrato a più riprese i sindacati, facendo il punto sulle principali criticità che interessano gli impianti di produzione, ed è stata definita una *road map* del confronto in corso con l'azienda. Il socio privato, dinanzi alla richiesta di impegno finanziario *pro quota*, ha detto con estrema chiarezza, nell'incontro di lunedì scorso a Palazzo Chigi, che non ha intenzione di immettere alcuna risorsa, persino per l'ipotesi in cui la sua quota, all'aumento del capitale sociale da parte della sola Invitalia, dovesse scendere al 34 ArcelorMittal si è dichiarata disponibile ad accettare di scendere in minoranza, ma non a contribuire finanziariamente in ragione della propria quota, scaricando l'intero onere finanziario sullo Stato, ma nel contempo reclamando il privilegio concesso negli originali patti tra gli azionisti, realizzati quando diedero vita alla società Acciaierie d'Italia, di condividere in ogni caso la *governance*, così da condizionare ogni ulteriore decisione, cosa che non è accettabile, né percorribile sia nella sostanza che alla luce dei vincoli europei sugli aiuti di Stato. Abbiamo quindi dato mandato ad Invitalia e al suo *team* di legali di esplorare ogni possibile conseguente soluzione. Sono queste ore decisive per garantire nell'immediato, in assenza di impegno del socio privato, la continuità della produzione e la salvaguardia dell'occupazione, nel periodo necessario a trovare altri investitori privati di natura industriale. Questa è la situazione che abbiamo davanti a noi, pregiudicata dalle decisioni assunte negli anni precedenti, nella scorsa legislatura. situazione a cui tutti insieme dobbiamo ora rimediare con la massima assunzione di responsabilità. Siamo consapevoli dell'importanza delle decisioni che dobbiamo assumere e quindi riteniamo importanti le indicazioni che le forze politiche vorranno esprimere anche in questa sede, anche nella seduta odierna. stato chiaro e mi attendo altrettanta chiarezza da parte vostra, nell'assoluto rispetto per quello che è il luogo sovrano della rappresentanza popolare, il nostro Parlamento.

*(IV-C-RE)*. Signor Ministro, l'ho ascoltata con grande attenzione perché l'acciaio - come ha detto del resto anche lei - è davvero una parte fondamentale della nostra economia. Noi siamo un grande Paese esportatore e praticamente l'acciaio è dappertutto. Se noi non abbiamo l'acciaio, la nostra capacità di vendere all'estero di fatto si azzera o viene colpita in misura significativa. L'acciaio è importante anche perché dà lavoro: l'acciaio è una filiera fondamentale del nostro Paese. Inoltre, sono importanti gli investitori internazionali. E il nostro atteggiamento rispetto a questo caso è fondamentale, perché la nostra capacità di attrarre investimenti internazionali - anche se lei parla di Stato stratega, signor Ministro, e si dichiara contro le multinazionali - sarebbe un vero problema. Noi dobbiamo essere capaci di dare messaggi coerenti per attrarre investimenti internazionali. Nei pochi minuti che ho naturalmente non posso ripercorrere la storia, dal 1965, dell'acciaieria di Taranto e non cadrò neanche nella ricostruzione delle colpe degli ultimi anni, anche se - secondo me - il momento in cui c'è stata quella gara è stato l'unico in cui c'è stata una visione. Ciò nonostante - a mio avviso - cambiare le carte in tavola, come si è fatto successivamente, è stata una di quelle mosse che certamente non ha creato fiducia né in quell'investitore internazionale, né in tutti gli altri investitori internazionali. La comunità del *business* - come lei sa - è una e globale e, se fai delle cose scorrette a un investitore internazionale, lo sanno tutti. Allora, visto che lei è qui e ho poco tempo, mi posso soltanto concentrare su quello che avete fatto voi in quattordici mesi. Ricordo, signor Ministro, che lei era qui un anno fa e ci ha detto grossomodo le stesse cose: ha detto che avrebbe fatto un piano strategico per la siderurgia, ma siamo qui un anno dopo e quel piano non l'abbiamo ancora visto. Lei viene a parlarci di acciaio *green*, ma io vorrei chiederle: signor Ministro, cos'è? Me lo spiega cos'è l'acciaio *green*? Come si fa, con quali soldi? Se oggi l'investitore privato dice di aver messo 2 miliardi nell'Ilva e che il socio pubblico non ha messo gli stessi soldi, io le chiedo: abbiamo i soldi per fare l'acciaio *green*?

per quanto stratega, signor Ministro, l'acciaio non lo sa produrre. Visto che il presidente Bernabè, ha già detto che se ne vuole andare nel mese di settembre e abbiamo fatto finta di niente, vorrei capire lei con quali professionalità

cioè lei si è fatto cogliere in castagna perché il socio privato è arrivato lì e ha detto che si sarebbe ritirato. Che conoscenza avete voi di quella società se davanti ad una decisione così enorme, voi, lo Stato, la Repubblica italiana, vi siete fatti prendere in castagna? Ma le preparate le riunioni? Ci sono dei momenti, dei tavoli? Oppure vogliamo dire che forse il socio privato si è trovato davanti a un Governo che aveva due linee? C'era infatti lei,

per quella fabbrica e per quella filiera. Lei vuole andare all'amministrazione straordinaria. Ma questo, Ministro, è un fallimento. Come comprerà le materie prime una volta che dichiara fallita l'azienda? Come pagherà le bollette? E dove troverà un socio privato che venga a lavorare in un'azienda dove gli impianti sono ancora sequestrati ed è fallita? Perché ci sarà un giudice, quella è una procedura concorsuale, non è mica un modo per lei per mettere un commissario amico suo e liberarsi del socio privato. Tutto questo mentre c'è un'enorme comunità che che aspetta di sapere qual è il suo destino. A Taranto ci sono infatti persone che vivono di cassa integrazione e che non hanno nessuna prospettiva di uscirne... ... il reddito di cittadinanza a 700 euro al mese e ci sono persone che stanno sostanzialmente nella stessa situazione perché finché non avranno una prospettiva, prenderanno la cassa integrazione come fosse un Concludo. La verità è che siamo davanti al vostro ennesimo disastro, non c'è una prospettiva e, come ha detto il capo di Federacciai se un socio privato arriverà, accadrà forse tra tre-quattro anni, ma a quel punto la fabbrica sarà probabilmente chiusa con buona pace dell'economia italiana.

senatore Magni.

bene a fare la cronistoria, ma ha saltato un problema. Prima ancora di Mittal c'era un signore che si chiamava Riva, che ha dimostrato l'incapacità del capitalismo italiano di gestire in modo corretto una grande azienda. A Taranto è infatti successo di tutto nella gestione Riva. Loro però hanno fatto molti soldi, questo sì. Quindi la prima logica è quella di ragionare se il mercato è in grado di rispondere. La stragrande maggioranza pensa che la regolazione venga data dal mercato, io penso che venga data dallo Stato.

Ci sono tre questioni fondamentali. La prima è salvaguardare l'occupazione. La seconda è affrontare il problema del risanamento e della bonifica, in particolare di tutta la città di Taranto, perché il lavoratore non può essere messo nella condizione

i lavoratori e i loro rappresentanti vi dicono che la risposta deve esserci oggi, perché sapete benissimo che il rischio è che domani quell'azienda chiuda. Questo è il dato. Ministro,

Io vorrei capire se lo Stato decide di utilizzare tutti i mezzi per riappropriarsi di questo bene generale, perché senza acciaio

Chiudere una fabbrica è successo a tutti. Io ho firmato la chiusura di una fabbrica, ma eravamo in una situazione diversa, in tempi diversi, in una Regione che non era la Puglia. Quindi, c'è il problema di salvaguardare totalmente l'occupazione,

Governo. Non voglio abbandonarmi alle polemiche e alla strumentalizzazione politica di queste ore che leggo anche sui giornali e sui quotidiani regionali del nostro territorio. Mi riferisco soprattutto a una strumentalizzazione politica

il socio di minoranza Mittal nelle condizioni di chiedere indennizzi al Governo italiano per i danni che ha creato in quel territorio. Ci troviamo quindi in una situazione veramente paradossale

non ha fornito alcuna soluzione ad un dramma che vede il Governo completamente assente. La solita politica del piagnisteo, la solita politica dello scaricabarile; c'è una visione strategica e non c'è nessuna prospettiva. Non ha dedicato neanche una parola al problema ambientale e sanitario; ripeto, neanche una parola. in questi giorni ARPA e ASL attestano il superamento dei limiti degli inquinanti consentiti. Una fabbrica che dopo oltre un anno ancora inquina nonostante le prescrizioni AIA, le migliori tecnologie e una produzione ai minimi termini. Fatta questa premessa, Ministro, lei ha millantato l'esistenza di un patto parasociale, così come tutte le forze di centrodestra hanno millantato l'esistenza di questo patto parasociale. Io la invito a fornirlo, dato che lei è Ministro, perché l'unica cosa che è pubblica, a disposizione e che esiste è un accordo tra Invitalia e ArcelorMittal. Questo accordo innanzitutto non era al ribasso nei confronti dei lavoratori e conteneva la soluzione al problema. infatti non abbiamo scelto di adottare la politica del piagnisteo in piena pandemia, ma siamo venuti in quest'Aula a dare soluzioni. Quali erano le soluzioni del Governo Conte II? Erano basate su due linee strategiche, due processi strategici: in il cambio di paradigma a livello industriale, con cicli produttivi completamente diversi. Sono questi i patti leonini che a voi non vanno bene, ossia diversificare l'assetto industriale del territorio? Questo è quello che abbiamo detto in quell'accordo: una diversificazione industriale e una prospettiva anche di riconversione economico-sociale e culturale del territorio con il cantiere Taranto. Cosa avete fatto voi in questi sedici mesi? Lei, signor Ministro, ha parlato di nulla, ma ha dimenticato di evidenziare che cosa avete fatto voi. Avete cancellato innanzitutto gli investimenti;

Avete anche fermato i progetti della transizione equa, pari a oltre 1 miliardo, per un totale di 2,2 miliardi. State cercando di fermare anche quel progetto di riconversione. Noi abbiamo rimediato quindi a una serie di errori del passato, commessi anche e soprattutto da chi è il principale artefice, con quella scelta di aver individuato Mittal come soggetto industriale credibile, l'aver voluto continuare il ciclo integrale e soprattutto - qui è l'errore che poi è all'origine dell'eventuale contenzioso - l'aver occultato in sede di gara che l'impianto è ancora sotto sequestro: questa è la madre di tutte le problematiche. Signor Ministro, avete reintrodotto lo scudo penale nella speranza di non nazionalizzare e sperando di trasferire a Mittal le responsabilità dell'investimento. Ora finalmente l'alibi è caduto, così come anche tutte le dicerie. Avete concesso un prestito di 680 milioni senza garanzie per l'indotto e senza tutele sull'ambiente. Vi state accingendo anche a confermare un riesame dell'AIA che prevede solo ed esclusivamente il ciclo a carbone per dodici anni, come lei oggi ha confermato: questa è una certezza che noi abbiamo. La seconda certezza è che oggi siamo in mezzo alla strada, perché Mittal vi ha chiuso le porte in faccia - questa è la realtà - e in questi sedici mesi non siete riusciti neanche a individuare un soggetto industriale privato credibile: questa è la più grande accusa che oggi le rivolgiamo. Noi, come forza politica che ha dato delle soluzioni in discontinuità rispetto al passato, con un nuovo paradigma basato sulla diversificazione industriale e sulla riconversione economico-sociale e culturale, continueremo a lottare a lottare per questo paradigma, per la chiusura delle fonti inquinanti e soprattutto per la stipula di un accordo di programma, che il territorio chiede con forza al fine di nazionalizzare l'impianto e definire risorse e tempi per le tutele ambientali, dei lavoratori e e dell'indotto. Signor Ministro, Governo, forze di maggioranza, il tempo è scaduto, il tempo delle chiacchiere è finito. Qui rischiamo una bomba sociale, dato che ci sono imprese dell'indotto non ricevono i giusti pagamenti, lavoratori che rischiano i licenziamenti, imprese di autotrasporto che da tempo rivendicano il pagamento delle fatture e sono state in sciopero per tutto il periodo natalizio. per non parlare poi delle altre problematiche della città, dall'arsenale militare dove non ci sono più commesse sulla cantieristica, ai progetti fermi del cantiere Taranto. Inoltre, vorrei anche evidenziare la problematica relativa al porto di Taranto, oltre 300 lavoratori da marzo saranno anche loro in mezzo alla strada. Se non è questa una bomba sociale, che si aggiunge a quella ambientale e sanitaria, ditemi voi come la possiamo qualificare.

a livello di azionariato ma anche possibilmente decisionale. Tuttavia, in questo difficile momento di passaggio della vicenda ex Ilva, coi suoi impatti economici, occupazionali e ambientali, ma anche sanitari, sanitari, con questo mio intervento desidero richiamare l'attenzione sua e del Governo su un paio di aspetti, che di certo saranno già stati alla vostra attenzione, ma purtroppo anche in passato sono spesso passati in secondo piano, o quantomeno non hanno avuto l'attenzione dovuta, nonostante le grida di allarme e di sofferenza che si sono levate dalle categorie produttive, dai lavoratori e soprattutto dai vari territori del nostro Paese che sono stati coinvolti. La vicenda Ilva, ora Acciaierie d'Italia, è di certo una questione il cui cuore batte a Taranto, in questa bellissima ma anche bistrattata città che ha pagato e sta pagando un conto salatissimo alla ragion di Stato. Non dimentichiamoci

Da sempre Ilva, ora Acciaierie d'Italia, rappresenta una rete di presenza industriale sull'intero territorio nazionale: pensiamo a Genova o a Novi Ligure, alla mia provincia di Cuneo, a Racconigi, rimanendo strettamente al Nord. Questi stabilimenti, tutti insieme, danno lavoro a circa 2.000 persone: 115 a Racconigi, a Legnaro 25, a Novi Ligure 650, a Marghera 50, a Genova 950, a Milano 220. se allarghiamo la visione, non possiamo dimenticare gli stabilimenti della già controllata Sanac Spa, coi suoi impianti a Massa, a Gattinara, a Vado Ligure, a Drogastu in Sardegna, che oggi occupano ancora oltre 260 lavoratori dipendenti. Questa realtà territoriali - non tarantine, ovviamente - danno indirettamente lavoro a decine, se non centinaia di imprese, creano occupazione, economia, ricchezza, una parte importante del prodotto interno lordo del nostro Paese. Ecco quindi, signor Ministro, perché reputo che questi aspetti territoriali non siano solo tarantini o pugliesi, ma che, sebbene siano forse aspetti minori, di certo non siano meno importanti e che vadano seguiti con la dovuta attenzione, preso atto del fatto che i Governi precedenti se l'hanno fatto lo hanno fatto in modo sicuramente non all'altezza della situazione. La vicenda Ilva, come ho detto, è una questione nazionale. Penso che il Governo comprenderà che essa va letta e seguita, come abbiamo detto, in tutte le sue articolazioni. È opportuno, poi, ricordare sempre come il caso dell'Ilva e delle sue controllate sia e resti anche una gigantesca vicenda - tra le più grandi, se non la più grande nella storia del nostro Paese

parliamo di uno stato passivo accertato, cioè di debiti verso terzi, di oltre 6 miliardi di euro, di cui, anche tolta la gigantesca pretesa di 3 miliardi di euro avanzata dal solo Comune di Taranto, e di circa un miliardo di debiti prededucibili dallo Stato per le varie manovre di sostegno all'amministrazione, almeno 2,5 miliardi sono i crediti. Verso chi? Tali crediti sono verso i fornitori, verso le imprese, verso i lavoratori che chissà se vedranno mai soddisfatte queste pretese, seppure parzialmente o seppure in modo idoneo. Parliamo di un totale di oltre 17.000 posizioni creditizie, che interessano 14.000 dipendenti, 2.500 fornitori, imprese grandi e piccole, artigiani, professionisti, cioè l'Italia che lavora, l'Italia che produce, che abbiamo il dovere e il diritto di difendere in quest'Aula ogni giorno. Queste persone e queste imprese pagano lo scotto di decisioni prese in tutt'altre sedi.

lei e soprattutto il Governo a vigilare affinché in questa ulteriore nuova fase - da quanto abbiamo ascoltato, le idee mi sembrano abbastanza chiare - che si andrà ad aprire, vengano tenuti nella dovuta attenzione tutti i territori e i tessuti economici ove siano presenti la filiera e gli stabilimenti dell'ex gruppo Ilva, affinché non andiamo a chiudere delle realtà che oggi invece hanno bisogno di essere sostenute

così che tutti coloro che hanno lavorato per queste imprese, che fino ad ora hanno già rimesso miliardi nella vicenda Ilva, possano avere questa attenzione e magari la soddisfazione delle loro ragioni creditizie, che in altre parole le ragioni dell'amministrazione

auspico che non si determinino per il futuro dei nuovi scenari e che non si profilino ulteriori sofferenze dei tessuti economici, perché partendo da Taranto a Cuneo, passando per Alessandria, da Genova fino a Cagliari, si possa trovare soddisfazione. È fondamentale agire con determinazione per restituire al Paese una visione futura - credo che su questo il Governo e il Ministro abbiano le idee molto chiare - di questo *asset*, che è un fiore all'occhiello del sistema industriale italiano

le Commissioni congiunte a Montecitorio, ripromettendoci reciprocamente di lasciare agli storici la ricostruzione non solo della vicenda dell'ex Ilva, ma anche della siderurgia italiana. Ma lei oggi ci è ricaduto; e ci è ricaduto con una serie di omissioni, le stesse omissioni che aveva fatto a Montecitorio. Siccome abbiamo solo cinque minuti - come ricordava il collega Magni - io oggi le parlerò di presente e di futuro, ricordando però all'Assemblea e lasciando agli atti del Parlamento che nella storia che abbiamo alle spalle (che è una lunga storia, signor Ministro, che riguarda lei come riguarda me, ma riguarda lei con i partiti a cui è appartenuto e riguarda me con il partito a cui sono appartenuto), c'è sempre stata una certezza: la destra è sempre stata dall'altra parte. Era dalla parte dei Riva e di chi inquinava quando noi ci battevamo per la decarbonizzazione. La destra è sempre stata dalla parte di chi

rischi di Taranto, passando per Genova, Novi Ligure e tutti gli stabilimenti che ha dimenticato e che ha omesso, anche nella ricostruzione rispetto al futuro - che avevamo la certezza che non solo la svolta *green* fosse possibile, ma che fare una battaglia in Europa sulla decarbonizzazione fosse centrale. Glielo dico, ministro Urso, perché lei non è stato il solo a non credere in quella svolta alcuni anni fa. È agli atti del Parlamento ma non ci torno. Parliamo di oggi. Parliamo di oggi. Lei di nuovo ci dice che l'acciaio primario si farà in un'unica acciaieria, che gli acciai speciali si faranno a Terni e le rotaie a Piombino, che poi forse ci sarà la svolta *green*, ma non capiamo in quale modo, e che vuole un aiuto da noi (ma noi su questo ci siamo sempre stati). Dimentica Genova. Voglio ricordarlo: Genova c'è, esiste, ed esiste Novi Ligure. Esistono dei presidi industriali che non vanno dimenticati. *(Applausi)*. Ma io voglio riportarla, signor Ministro, sulle sue omissioni. ha completamente dimenticato di parlarci del *memorandum* firmato dal ministro Fitto e ha completamente dimenticato di dirci cosa c'era dentro questa lettera, che noi abbiamo potuto leggere solo qualche giorno fa. fa. Mittal scrive ad un certo punto non al Ministro delle imprese, ma al Ministro degli affari europei, dicendo di aver inviato un piano industriale con una serie di prerequisiti. Ma lei era al corrente che c'era un piano industriale? Non lo sapevano i lavoratori, non lo sapeva Invitalia, non lo sapeva il Parlamento, non lo sapeva nessuno. Glielo chiedo ancora oggi: cosa c'era nel *memorandum* sottoscritto dal ministro Fitto a sua insaputa e a insaputa del ministro Giorgetti? *(Applausi)*. E cosa c'è in questo piano industriale?

entrate subito nel capitale. Mittal ha comprato le quote di mercato e chi le parla si è espresso quando i Governi della propria parte politica stavano facendo quella scelta, perché è stata una scelta bizzarra vendere in conto affitti. Penso che, nella storia industriale del globo, una cosa eccezionale. Ma ce le siamo già dette queste cose; parliamo di presente e soprattutto di futuro. Questo pomeriggio, per la prima volta, assumervi delle responsabilità. Dovete dire con chiarezza ai lavoratori che incontrate quali scelte farete, senza fare giri particolari di parole, perché non ci sono solo 20.000 20.000 lavoratori (10.000 dell'ex Ilva e 10.000 dell'indotto), ma c'è l'intero sistema siderurgico italiano che aspetta una risposta. Ministro Urso, finora abbiamo sentito - e qui ce le ha confermate ipotesi contrastanti e incompatibili tra loro: nazionalizzazione, liquidazione della società, attivazione di un'ennesima amministrazione straordinaria. Sintomi, a nostro avviso, di una mancanza di chiarezza e di visione che rischia di fare solo gli interessi di un soggetto privato che ha spostato gli interessi, per sua stessa ammissione, fuori dall'Italia e fuori dall'Europa. Se amministrazione straordinaria deve essere, lo decidete voi e ve ne assumete la responsabilità: l'amministrazione straordinaria va fatta con almeno un miliardo di fondo speciale immediato per garantire l'indotto, per garantire i lavoratori e per garantire un passaggio senza traumi. Se così non dovesse essere, vi assumete la responsabilità di sostituire il socio privato, di ricorrere alle tante eccellenze che abbiamo ancora in Italia. Ricordo a tutti noi, perché le analisi le abbia fatte il Partito Democratico, che World Steel Association nell'ultimo *outlook* di quest'anno, ci dice che in Italia nel 2024

Stiamo parlando di prospettive industriali che abbiamo il dovere di accompagnare, di garantire e, laddove non fossero pronti i privati, di intervenire guidando questo processo. L'unica cosa che non possiamo più permetterci, signor Presidente, sono le vostre omissioni e le vostre divisioni. Finora, in quindici mesi, abbiamo avuto da tre Ministri

signor Ministro, la ringrazio da pugliese, non solo per l'esaustività della sua relazione, ma soprattutto per l'impegno e il lavoro che fin dal primo giorno del suo insediamento e dell'insediamento del governo Meloni avete profuso per poter dare una soluzione a un altro fardello che abbiamo ereditato e che hanno lasciato sulle nostre spalle. Oggi ho sentito diverse chiacchiere e accuse, ma non siamo stati noi quelli che calcavano le scene elettorali a Taranto per farne culla della cultura della morte e aumentare i consensi elettorali, né siamo stati noi quelli che calcavano le scene elettorali a Taranto per costruire palcoscenici di illusioni, per trasformare l'ex Ilva in parchi archeologici, tecnologici, acquatici e non si sa più che cosa. Non siamo stati noi quelli che hanno scelto il socio privato. Non siamo stati noi quelli che hanno tolto lo scudo penale che era nell'accordo contrattuale e che ha posto il nostro Paese, il nostro Stato, in una posizione minoritaria di forza rispetto agli impegni che erano contenuti nell'accordo tra le due parti. Non siamo stati noi quelli che si sono divisi; noi siamo uniti, ma ricordo che le divisioni erano nel Partito Democratico, durante il Governo Renzi, con Calenda e Gentiloni che controbattevano con il presidente Emiliano. Le divisioni erano nel MoVimento 5 Stelle, quando la senatrice Lezzi controbatteva con il Governo Conte per rimuovere lo scudo penale, riuscendoci Quindi, la regola di uno vale uno in quel momento non è valsa, perché la senatrice Lezzi è valsa molto di più dell'uno, anzi di tanti. Si dice che lei, Ministro, non ha le idee chiare. Caro Ministro, io invece dico che le sue idee non solo sono chiare, ma sono anche giuste. Come si può venire qui, all'esito di questa tragedia, e avere una soluzione pronta? Non farebbe il bene dell'Italia. Ha fatto bene lei a vagliare tre ipotesi di soluzione e questo è il punto di forza della sua informativa: lei ci sta dicendo che vaglierà le diverse possibilità e le diverse soluzioni, scegliendo quella più opportuna, più idonea e più utile al nostro Paese, alla maggioranza degli degli italiani e alla nostra Puglia. Anche sul passaggio dell'ambiente, colgo le parole del Ministro. ha parlato di senso di responsabilità, conseguenze sulla salute, processo di riconversione ambientale; sono parole che vanno nella direzione giusta perché, caro senatore Boccia, mi rivolgo a lei tramite il Presidente, noi siamo per la contemperanza tra valori di pari rango costituzionale. Siamo per l'occupazione e il lavoro, per la tutela della salute e dell'ambiente. Siamo per questo dentro il piano articolato che ha prospettato il ministro Urso poco fa. Siamo dentro una responsabilità che ci pone nella condizione di poter offrire una speranza concreta e non un'illusione (non l'illusione dei parchi acquatici, dei parchi tecnologici, dei parchi per la mitilicoltura); la speranza di una rinascita di questo sviluppo industriale in un settore strategico del nostro Paese che lo pone a livello europeo. Abbiamo infatti ben presente cosa significa questo stabilimento per il nostro Paese: PIL,

Saremo sempre con lei e con il Governo perché abbiamo fiducia nel Governo e abbiamo fiducia nelle sue parole e su quanto lei ci ha detto. Noi ci crediamo, signor signor Ministro, ci crediamo insieme a lei. Noi ci impegniamo a ricostruire su impianti *green*; sì, ci impegniamo insieme a lei. Abbiamo fiducia in lei, abbiamo fiducia nel Governo, vada avanti, noi siamo e saremo con lei.

chiede di intervenire ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Regolamento, che prevede che un Ministro di un precedente Governo possa chiedere la parola qualora ci sia stato un riferimento a provvedimenti di quel Governo. Siccome, obiettivamente, qualche riferimento c'è stato, non ho difficoltà

Ministro. Anche oggi accetto visioni e proposte diverse; ne ho sentite poche invero nella relazione, ma non voglio entrare nel merito politico del dibattito sulla relazione del Ministro, che anzi ringrazio per essere venuto oggi in Assemblea. Entro nel merito invece su alcune affermazioni che sono state in parte omissive e in parte non veritiere rispetto all'operato dei governi di cui ho fatto parte. Mi soffermo su tre elementi in particolare. Il primo elemento è il tema dell'esimente penale. Il Ministro è stato omissivo e il senatore Zullo è intervenuto, per il suo tramite, Presidente, altrettanto. L'offerta fatta da Mittal era un'offerta incondizionata e non conteneva riferimenti alla presenza di una esimente penale e non potrebbe essere diversamente dato che non ci può essere un accordo che preveda un blocco un blocco dell'azione legislativa libera delle Aule parlamentari o della decretazione di un Governo. Quindi non ci può essere un accordo che preveda il mantenimento di una norma. *(Applausi)*. Questo è il primo elemento.

a dimostrazione che quello sarà stato forse un pretesto, ma certamente non un elemento che in qualsiasi aula di tribunale, in caso di causa per il recesso unilaterale di Mittal, avrebbe avuto alcun effetto sull'esito del contenzioso. Sono stati citati i patti parasociali, che però sono un elemento di diritto privato; non esiste un Governo che possa sottoscrivere patti parasociali. È falso sostenere che esistano patti parasociali segreti; esiste un accordo di coinvestimento che il Governo ha autorizzato i commissari

Il tema della *governance* prevede inizialmente, con l'ingresso al 38 per cento di Invitalia, la possibilità per il socio privato di nominare l'amministratore delegato, per il socio pubblico di nominare il presidente, un pari numero di consiglieri e il presidente del collegio sindacale di nomina del socio pubblico, con le deleghe che il Ministro ha citato e con il gradimento reciproco (che è previsto). Questo è stato citato dal Ministro come uno degli elementi del patto leonino, perché diamo tutto in mano al socio privato. Con l'aumento del capitale di Invitalia al 60 per cento si invertono le potenzialità di nomina, quindi se prima era leonino per noi, dopo diventa leonino per il socio privato, perché questo è previsto nell'accordo di coinvestimento. Su questo elemento il Ministro

il cantiere Taranto, con investimenti privati, come ad esempio quelli del Gruppo Ferretti, e abbiamo inserito una penale per recesso immotivato da 500 milioni di euro, come lei ben sa, cosa che non era prevista precedentemente. Abbiamo quindi migliorato enormemente l'accordo iniziale sottoscritto nel 2017. inoltre lasciato una prospettiva industriale. Io mi auguro e confido che questo Governo abbia una prospettiva industriale. Al momento, in tutti i provvedimenti che abbiamo analizzato in queste Aule, di progetto industriale per il Paese non c'è assolutamente traccia.

finestra") sulla candidatura della cucina italiana quale bene patrimonio dell'umanità UNESCO, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si è deciso di proporre la candidatura ufficiale della cucina italiana quale bene patrimonio dell'umanità UNESCO per il 2023. La commissione nazionale ha già approvato all'unanimità la proposta, che passa ora all'esame del comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale e materiale. Il *dossier* poi verrà trasmesso al Ministero degli affari esteri e all'UNESCO, dove inizierà l'*iter* di valutazione. La decisione è attesa per il 2025. È assodato come la nostra cucina sia mosaico di tradizioni che riflette la diversità bioculturale del Paese. Intorno alla nostra cucina italiana si racchiude un insieme di valori che, muovendo dal variegato patrimonio enogastronomico, ricomprende aspetti che interessano la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese che, trovando concretezza nei tanti

circa 60 milioni, ma anche i 70 milioni che vivono al di fuori del nostro Paese, e che amano mantenere vive le tradizioni alimentari italiane, e anche tutti gli stranieri che amano la nostra cucina e il nostro Paese. Ad oggi fanno parte del patrimonio immateriale UNESCO le cucine messicana, francese, giapponese e coreana. Senza nulla togliere a queste realtà culinarie, a maggior ragione la nostra cucina italiana deve prendere il posto che le compete, visto l'enorme apprezzamento di cui gode a livello internazionale. La candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'umanità è poi la risposta a chi invece vorrebbe imporci una dieta globale fondata su insetti e cibi sintetici, senza alcun legame con i nostri territori; un annuncio che arriva con il *record* storico realizzato dalle esportazioni agroalimentari *made in Italy* nel mondo, per un valore di di 60,7 miliardi. Dato che il Governo ha avuto la grande intuizione di abbinare la forte capacità attrattiva della nostra lunga tradizione enogastronomica a quella dell'immenso patrimonio culturale italiano, quali iniziative ed eventi saranno portati per presentare la candidatura della cucina italiana quale patrimonio dell'umanità in Italia e all'estero e per promuovere l'idea della qualità del vivere italiano, che è fatto di arte, di cultura, di paesaggi, al fine di dare ancora maggior lustro alla cultura enogastronomica e alla dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come lo stile di vita più sano al mondo?

senatrice Minasi per avermi interrogato su questo punto. Le rispondo innanzitutto con un richiamo chiaro alla nozione di immaterialità. L'UNESCO da qualche anno ha riconosciuto che non esistono soltanto dei valori materiali, cioè delle cose tangibili (Pompei, il Colosseo, l'Arena di Verona), cioè dei siti che possiamo guardare e ammirare nella loro materialità, ma ci sono anche, parimenti importanti, non meno importanti, le immaterialità, cioè quell'insieme di tradizioni, di arti, di mestieri e di saper fare che si tramanda di generazione in generazione e che è indubbiamente un valore e una tradizione della nostra Nazione che dobbiamo preservare e tutelare coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione. Pertanto, immaterialità è tradizione, creatività, conoscenza ed è la componente culturale in cui il nostro popolo si identifica. Credo che l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale della cucina italiana sia quasi un atto dovuto; come ha ricordato l'interrogante, ne fanno già parte la cucina francese, la cucina coreana, la cucina giapponese, verso le quali io ho il massimo rispetto e apprezzamento, ma è singolare che la cucina italiana non ne faccia parte.

di tanti territori e di tante esperienze regionali: non c'è località, anche piccola, del nostro territorio nazionale che non abbia un qualcosa, una pietanza da proporre frutto di una lunga tradizione. Si tratta, pertanto, di una grande operazione di sistema. Del resto, la qualità della vita delle persone è data da una sanità efficiente, da un contesto urbano efficiente, dai trasporti, dalla mobilità, dalla scuola, dall'istruzione, dalla cultura.

chiaro riferimento anche alla qualità del cibo. Noi siamo quindi impegnati in questa operazione di sistema. Stiamo creando una serie di manifestazioni in tutte le Regioni italiane: una c'è stata a Pompei, ma le faremo anche in Lombardia, in Veneto, in Sicilia, in Calabria; ovunque noi cercheremo di rappresentare tutto ciò, perché crediamo che possa essere un fattore positivo.

alla cucina italiana il titolo di patrimonio immateriale dell'UNESCO significa anche alimentare l'orgoglio nazionale e il senso di appartenenza degli italiani al loro Paese e mi riferisco sia a chi oggi risiede in Italia, sia a chi - come ho già detto prima - vive all'estero ma continua a a mantenere forte un legame con la Patria. Anzi, forse la cucina italiana è proprio uno dei principali collanti che unisce tutti noi connazionali. Io in particolare, soprattutto da calabrese, posso certamente testimoniare quanto la cucina italiana sia un pezzo preponderante della stessa vita familiare e sociale, quanto scandisca la vita familiare e la socialità sia nel quotidiano che nelle occasioni speciali. Inoltre, in conclusione, ricordo e sottolineo anche come la cucina italiana possa - come ha già detto il signor Ministro prima - contare su una varietà enorme e difficilmente enumerabile di ingredienti tipici unici dei nostri territori e soprattutto genuini, che appunto la differenziano dal resto del mondo e la rendono davvero rendono davvero esclusiva, tanto da essere la più ricercata. Bisogna pertanto continuare a investire, ma soprattutto a tutelare l'unicità del nostro comparto agroalimentare e l'ottenimento del riconoscimento UNESCO certamente rappresenterà uno strumento preziosissimo in questa direzione.

ha ottenuto riconoscimenti positivi dalle principali agenzie di *rating*. Tali riconoscimenti sono suffragati peraltro dai dati positivi dell'Istat in merito al tasso di occupazione, alla crescita del reddito e del potere d'acquisto delle famiglie e al calo della pressione fiscale. Grazie al contributo fattivo e al senso di responsabilità dei parlamentari di maggioranza, inoltre, con la legge di bilancio per il 2024 il Governo ha fornito diverse risposte alle imprese, dimostrando di mantenere fede al programma presentato agli elettori. La legge di bilancio ha dovuto anche tener conto delle sfide di transizione *green* e digitale in atto, al fine di salvaguardare le imprese italiane in questa delicata fase. Grazie all'operato del Governo Meloni l'Italia, infatti, sta portando in Europa una filosofia capace di tenere insieme transizione *green* e tutela del nostro sistema produttivo. Una prova recente di ciò si è avuta con il piano Transizione 5.0, approvato dalla Commissione europea già nel novembre 2023 nell'ambito del REPower EU, che rappresenterebbe l'evoluzione del piano Transizione 4.0. Questo piano servirà a rendere più competitive le imprese italiane in Europa e nel mondo, a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e al contempo a garantire il rispetto degli impegni europei sulla transizione verde in forme che possono risultare sostenibili per le imprese del nostro Paese. Pertanto, al di là di talune polemiche strumentali, Ministro, dalla legge di bilancio e dal piano Transizione 5.0 emerge, in linea generale, la volontà dell'Esecutivo di essere al fianco del mondo produttivo italiano nel cammino verso una transizione verde e digitale guidata dalla ragionevolezza e non dall'ideologia. Si chiede, quindi, di sapere quali misure nello specifico il Governo abbia previsto a favore delle imprese e quale sia lo stato di attuazione del piano di Transizione 5.0.

ha agito su due piani, come se fossero due binari, per recuperare risorse utili alle imprese in questa importante, significativa sfida alla duplice transizione. Sul piano del bilancio nazionale, siamo riusciti a recuperare 5,3 miliardi in più per le imprese; un miliardo in più per i contratti di sviluppo;

arrivando a una disponibilità di 3 miliardi per i fondi e per le imprese che utilizzano i progetti IPCEI; più altre risorse come il finanziamento della Sabatini e il Fondo per la sostenibilità. In totale, In totale, parliamo di 5,3 miliardi, comprese le risorse per le ZES nella manovra di bilancio. Un'altra manovra di fatto l'abbiamo fatta in sede europea, con la revisione del PNRR, attraverso il capitolo REPower EU. E, attraverso questa manovra aggiuntiva che abbiamo fatto in Europa, abbiamo destinato 14 miliardi alle imprese, quasi 10 miliardi in più al mio Dicastero, 2,8 miliardi per le imprese agricole (Ministero dell'agricoltura) per l'efficientamento energetico e quasi due miliardi per le imprese che realizzeranno la connettività (gasdotti e reti elettriche) che sono a controllo pubblico. Ma venendo al mio Dicastero, quasi 10 miliardi si aggiungono a queste cifre e a quanto già contenuto nel bilancio nazionale. Questo significa che dai prossimi mesi saranno disponibili tre miliardi e mezzo miliardi e mezzo dai fondi del REPower EU e un miliardo dai fondi nazionali) per i contratti di sviluppo, cioè per quelle imprese che investiranno in siti produttivi, tanto più per tecnologia *green* e digitale. E soprattutto saranno disponibili quasi 13 miliardi per il piano Transizione 5.0: milioni dai fondi europei REPower EU e 6 miliardi e 400 milioni che erano già nel bilancio nazionale. In totale, quasi 13 miliardi per il piano Transizione 5.0, che presenteremo in decreto-legge tra poche settimane, in modo da renderlo immediatamente operativo, tanto più che abbiamo già preparato i decreti attuativi. In questo caso significa innovazione digitale per le imprese, in un programma complessivo che può e deve contenere anche l'efficientamento energetico per la riduzione del consumo energetico delle imprese attraverso impianti di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo. In totale sono 13 miliardi. Il 10 per cento potrà essere destinato alla formazione, cosa che le imprese ci chiedevano molto, per poter utilizzare le nuove tecnologie digitali e le nuove tecnologie *green*. In questo modo abbiamo messo in campo riforme e risorse sufficienti per accompagnare e sostenere lo sviluppo delle nostre imprese, sia di quelle che vogliono realizzare nuovi impianti produttivi (tre miliardi e mezzo in contratti di sviluppo), sia di quelle che vogliono innovare i propri macchinari (Transizione 5.0, che ingloba anche Industria 4.0),

testimonia, c'è l'andamento dei mercati finanziari, che vede la Borsa di Milano avere progressioni importanti mai viste negli ultimi anni. Come ho detto nell'*incipit* dell'interrogazione, ci sono il giudizio delle agenzie di *rating* e anche l'andamento del nostro *spread*, che oggi ci vede ampiamente al di sotto dei dati dei precedenti Governi. Quindi, grazie, Ministro, per quello che sta facendo.

Grazie, Presidente, lei è molto gentile. Spero di poterci arrivare, a differenza di altri a cui è precluso in partenza. il 31 dicembre il Presidente della Repubblica fa un grande discorso. Tutti lo applaudiamo e la Presidente del Consiglio per prima gli fa la telefonata di rito. Nel discorso del Presidente della Repubblica c'è un passaggio sull'utilizzo delle armi, sul rischio della diffusione dell'utilizzo delle armi. Tutta Italia applaude, a cominciare dalle forze politiche di maggioranza. Passano quattro ore e dal Quirinale dobbiamo andare nella provincia di Biella, in un Comune di 99 abitanti, dove si svolge un veglione organizzato dal suo Sottosegretario alla giustizia - Sottosegretario di tutti,

ed è l'argomento della richiesta che le facciamo nell'interrogazione: quanti erano gli agenti della Polizia penitenziaria? Chi di noi si avvale del prezioso servizio degli agenti, delle donne e degli uomini della scorta, sa quanto sono bravi, sono dei professionisti. Ma non vanno a cena insieme: proteggono la personalità a cui sono assegnati. Invece in questo caso c'è un clima di familiarità, anche perché il capo scorta è un collega politico, sindacalista e amico. È una cosa un po' strana, non ha molti precedenti nella storia repubblicana. Nel corso di quel cenone accade a un certo punto che arriva un deputato dello stesso partito, Fratelli d'Italia, un vostro collega, che tira fuori una pistola. Forse non aveva fatto in tempo ad ascoltare il messaggio del Presidente della Repubblica, ma non ci sono battute da fare, pensando che in quella sala c'erano anche dei bambini. E tirando fuori la pistola, come nelle peggiori sceneggiature, a un certo punto la pistola esplode un colpo, ma il Sottosegretario non è in quella sala, perché è uscito.

va a 400 metri di distanza e tutti gli agenti di polizia penitenziaria - noi li paghiamo per proteggere il Sottosegretario - non lo seguono, ma rimangono a gozzovigliare, o più banalmente a controllare l'arma che esplode un colpo. Non si capisce chi sia stato, perché nessuno ha visto Pozzolo, cioè il deputato, che continua a negare di essere stato. Non si capisce chi sia stato, perché non c'è una testimonianza univoca. E il Sottosegretario non ravvisa il pudore istituzionale di dire che intanto rimette la delega alla polizia penitenziaria, se non addirittura è chiaro che qualcuno sta mentendo agli italiani e c'è da augurare che non abbia mentito a lei nella relazione. Le domando: lei è in grado di stabilire quello che è successo? Io ho messo la vicenda in modo ironico, parla di una pistola che ha colpito un uomo e poteva ucciderlo in una sala piena di bambini. Se questo vi sembra un comportamento degno di una persona che riveste il ruolo di deputato, evidentemente abbiamo due concetti diversi di dignità.

Onorevolissimo collega Renzi, mi permetto di risponderle da ex magistrato che è stato sottoposto a tutela negli anni Ottanta, quando indagava sulle Brigate Rosse. La tutela è stata rinnovata successivamente, vari anni, quando mi sono occupato di tangentopoli, di mafia e da ultimo del Mose e, quindi, so come funziona. Esiste una forma di tutela esterna, che è quella che si occupa della garanzia del tutelato per quanto riguarda gli ambienti circostanti; una volta che questa è stata assicurata, esiste una tutela interna: se il tutelato rimane in un ambiente chiuso, deve essere accompagnato da chi deve assicurarne la tutela. Quindi, non vi è nulla di scandaloso se a una manifestazione conviviale partecipano anche le persone che devono tutelare chi partecipa a quella situazione conviviale. Per quanto riguarda la scelta delle persone di tutela, posso assicurare che essa è individuata - cito solamente i regolamenti - dal provveditorato regionale competente e non è minimamente scelta - questo lo dico anche a titolo personale - dall'autorità che è protetta: si chiama «nota personalità» o «Monza 500» nell'ambito delle tutele. può e non deve esservi alcun sospetto di contiguità partitica, politica, ideologica o altro tra gli uni e gli altri. Poi, naturalmente, la forma della partecipazione ad attività conviviali, compreso chi viene invitato, è oggetto che non può essere trattato qui dal Ministro della giustizia, perché è discrezionale ed è deputato alla libertà personale di chi organizza la convivialità. Da ultimo, sull'episodio, vorrei parlare da magistrato e non posso. Dovendo parlare da Ministro, non posso che inchinarmi di fronte a quello che è il segreto istruttorio. Sono in corso delle indagini, sarebbe improprio, forse addirittura - come si è sentito dire - delittuoso se io qui rivelassi delle cose, ammesso che le sapessi. Se devo dire la verità, non le so, perché il segreto istruttorio è stato - per fortuna - doverosamente tutelato. Va da sé che, nel momento in cui un domani dovessero emergere da parte della magistratura delle ricostruzioni adeguate e obiettive, sarei il primo a riferirle davanti a questo onorevole consesso. di tanto non posso dire perché - ripeto - noi ci inchiniamo di fronte a quelle che sono l'autonomia e la tanto decantata indipendenza della magistratura. Se posso citare un suo illustre concittadino, «e questo fia suggel ch'ogn'omo sganni».

di fronte a scene di assoluta incapacità istituzionale come sono quelle del suo Sottosegretario e del suo compagno Pozzolo. Mi spiego:

il giudizio politico nell'utilizzazione della scorta da parte del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e nelle responsabilità atroci di portare armi da fuoco in una sala dove ci sono bambini, nella ricostruzione che è chiaramente fallace. è stato più volte sotto tutela per cause molto serie. Lei non si è mai fatto 400 metri a piedi nella notte da solo. Qui non si può discutere se il capo scorta,

ma visto che c'è tutta quella allegra combriccola, uno che esca con il Sottosegretario a controllare dove sta andando nel pieno della notte, vogliamo considerarla come un'ipotesi che abbia un senso oppure vogliamo giustificare il fatto che il capo scorta rimanga nella sala mentre il Sottosegretario non c'è? questo è il mondo all'incontrario e che ci state prendendo per pazzi? Aggiungo, signor Ministro, che le ricostruzioni non tornano. A me non interessano l'indagine che farà il pubblico ministero e il giudizio che darà un giudice. Non mi interessa che vi sia un colpevole giudiziariamente. Figuriamoci se io posso essere interessato a questo. Io ritengo, e - tramite la Presidenza - lo dico ai colleghi e amici della maggioranza, che questa vicenda denoti una incultura istituzionale spaventosa, un utilizzo proprietario della polizia penitenziaria e una reticenza omertosa di fronte alla verità. La notte di Capodanno avete toccato il fondo:

avranno le loro sedi. La nostra è un'interrogazione sulla responsabilità politica, sul ruolo della politica, sulle posture istituzionali e sulla incompatibilità politica. Quando ci riferiamo a questo, parlare di opportunità è davvero troppo poco. I fatti che si sono verificati durante il veglione a Rosazza Molti aspetti, stando anche agli articoli di giornale che si stanno susseguendo e dalle notizie che apprendiamo dagli organi di stampa, sono ancora molto da chiarire e destano, a dir poco, perplessità sul piano politico e istituzionale. Consideriamo intanto il contesto: risulterebbe che diversi agenti della Polizia penitenziaria erano presenti alla festa insieme alle loro famiglie. Risulta che il capo della scorta, l'ispettore capo Pablito Morello, agente della Polizia penitenziaria, sia stato scelto personalmente dal Sottosegretario. Risulta che l'ispettore capo Morello condivida una comune militanza politica con il Sottosegretario. Perché tutto questo ha una sua rilevanza?

Uno dei tavoli del ristorante che ha ospitato l'evento è stato riservato alla Polizia penitenziaria. In quella occasione c'è stata una dimostrazione di solidarietà verso il sottosegretario Delmastro, perché c'era uno striscione, appunto appunto della Polizia penitenziaria, dove si diceva: siamo tutti Delmastro. Alcuni agenti della Polizia penitenziaria hanno sfilato tra i tavoli indossando una maglietta con scritto: «Anche io sono Delmastro». fin superfluo ricordare che, tra l'altro, il Sottosegretario si è reso responsabile del fatto di aver rivelato a un collega di partito il contenuto di documenti che non erano divulgabili. A noi non interessa assolutamente la vicenda giudiziaria. Resta il fatto, inoppugnabile e ormai pacifico, che non erano divulgabili. E resta ancora un mistero, signor Ministro, cosa abbia spinto lei, appunto un galantuomo, ad affermare nelle Aule del Parlamento esattamente il contrario. Ancora, ci sono diverse vicende che hanno interessato l'istituto penitenziario di Biella, che sono state oggetto di inchiesta della magistratura. Diversi agenti sono stati sottoposti a indagini per reato di tortura, sospesi dal servizio e poi reintegrati. È stato oggetto di una di una nostra interrogazione il fatto che vi sia stata una grigliata alla fine di luglio, presente sempre il sottosegretario Delmastro e presenti quegli agenti reintegrati, dove si sarebbero celebrati dei brindisi per l'abolizione del reato di tortura. Ancora, sempre

Il Ministro della giustizia non ritiene opportuno chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra il sottosegretario Delmastro e alcuni settori della Polizia penitenziaria vicini al suo partito? Chiarire, cioè, se questi rapporti non abbiano creato una sovrapposizione tra il ruolo istituzionale che la delega assegna al sottosegretario Delmastro e l'attività di propaganda di partito. Infine, tutti i fatti ricordati fanno ritenere ancora compatibile l'esercizio di una delega così delicata in capo all'onorevole Delmastro? Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, stiamo parlando di politica, di ruolo e postura istituzionale, elementi imprescindibili quando, come avviene spesso, in quest'Aula e pubblicamente, ci si appella alla centralità della politica, intestandosi la sua presunta ricomparsa in queste Aule.

dalla stessa sua esposizione, che è giustamente molto limitata dall'uso del condizionale, certe cose non si sanno. Lei ha usato i tempi verbali: sarebbero, ci sarebbe stata, sarebbe avvenuto. Sono, cioè, notizie che si hanno attraverso la stampa, di cui noi non abbiamo né certezze né plausibilità, visto che molto spesso, anzi frequentemente, purtroppo oggi le *fake news* sono la regola più che l'eccezione. È per questo che ritorno a dire quello che ho detto prima. Ella ha citato anche l'episodio della divulgazione di segreti. Vi è una indagine in corso; è stata chiesta una archiviazione ed è stata imposta una imputazione coatta. Vedremo come andrà a finire Qui c'è un'indagine in corso. Noi non possiamo, in questa sede, introdurre il condizionale, introdurre l'ipotetico. Aspettiamo che sia la magistratura ad accertare cosa sia avvenuto realmente quella sera e poi non ci sottrarremo alle risposte anche politiche che dovremo dare. Per quanto riguarda i rapporti tra il Sottosegretario e la Polizia penitenziaria, il Sottosegretario ha la delega.

Vorrei citare una circostanza politica importante: in occasione di una formale riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, celebrata il 16 novembre, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e quindi tutte le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, hanno pubblicamente manifestato vivo e sincero apprezzamento per l'impegno che è stato profuso dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove *(Applausi)*. Se la gratitudine

Chi comanda la vita del tutelato è il responsabile della scorta. Fa una vita monacale, come la faccio io, ma deve farla perché questo è il suo impegno. Vorrei però che molti, anche rappresentanti di Governi precedenti e anche ex Ministri

Io temo che questo sia accaduto nel passato; con me non avviene. Se sul proprio onore tutti i presenti sono disposti ad affermarlo, allora sarò ben lieto di prenderne atto. Per quanto riguarda poi - ripeto ancora una volta - le frequentazioni personali di quella determinata cena, si tratta di una scelta discrezionale che esula dalle competenze del Ministro della giustizia.

Anna Rossomando ha detto molto bene - chiarezza sui rapporti ambigui tra il sottosegretario Delmastro, settori della Polizia penitenziaria e i suoi agenti di scorta, anche suoi stretti sodali di partito. Ma lei non ha risposto. Chiediamo chiarezza sulla partecipazione di Delmastro a quelle grigliate, in carcere a Biella, mentre le carceri italiane scoppiano, *(Applausi)* mentre ogni giorno un detenuto si toglie la vita e mentre in quel carcere sono avvenuti fatti gravi, oggetto di provvedimenti della magistratura. Lei ha glissato e continua, Ministro, a coprire questo Sottosegretario inadeguato - altro che consenso - come quando lo stesso aveva prodotto carte a divulgazione limitata - sue parole, Ministro - in quest'Aula a un suo compagno di partito per colpire l'opposizione e per questo è stato rinviato a giudizio; un Sottosegretario che organizza veglioni con la scorta con bambini, ai quali va anche un deputato del suo partito, con una pistola che fa fuoco e ferisce una persona. È una storiaccia. Farà chiarezza la magistratura, visto che nessuno di voi vuole spiegare come è andata davvero e perché un parlamentare del vostro partito gira armato. Ho finito, Presidente. Delmastro dovrebbe dimettersi, altrimenti dovrebbe essere la presidente Meloni a farlo dimettere, a togliergli deleghe che non può mantenere. La nostra Segretaria ieri ha detto che Meloni è prigioniera del proprio passato. Aggiungo che è prigioniera anche del proprio presente, di alcuni sodali di partito inadeguati *(Applausi)*, che non sanno cosa sia il senso dello Stato e questo, Ministro, mi dispiace dirle che, insieme alla sua complice inerzia, carica anche lei e il Governo di una grave responsabilità.

ministro Nordio, i toni del mio intervento saranno meno polemici rispetto a quelli dei colleghi che mi hanno preceduto. Signor Presidente,

Ministro e stiamo affrontando temi molto importanti come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la stretta sulle intercettazioni,

con un tono marcatamente garantista, che è proprio quello che lei ha sempre manifestato in tutta la sua esperienza, prima di magistrato e poi di politico. Le chiedo altresì, signor Ministro, di illustrarci le ulteriori iniziative del Governo, perché il tema della riforma giustizia è molto ampio. Mi permetto di sollecitare una sua risposta su due temi che mi stanno particolarmente a cuore, il primo dei quali è la stretta sull'utilizzo del *trojan*, questo mezzo così intrusivo e pervasivo che indaga le vite delle persone. Lei, Ministro, sa bene che io personalmente e l'intero mio partito su questo tema ci siamo impegnati e vi sono state delle iniziative legislative. In particolare, in occasione della discussione alla Camera del decreto-legge *omnibus* sulla giustizia, abbiamo ritenuto di ritirare tutte le nostre iniziative in attesa di un un provvedimento da parte del Governo. So che lei sta lavorando su questo tema e so che c'è una commissione ministeriale in corso. Il tema è complicato e delicato, però vorrei che oggi lei ci dicesse quali saranno i tempi affinché questo argomento possa arrivare all'esame dell'Assemblea. secondo tema che sottopongo alla sua riflessione, che pure è una delle questioni che mi stanno a cuore e che sono state oggetto di mie iniziative anche nella precedente esperienza di consigliere superiore della magistratura. Mi riferisco all'utilizzo disinvolto dei *social media* da parte dei magistrati. Ho sempre detto che il magistrato deve avere un particolare contegno che ne garantisce l'autorevolezza e la terzietà e che quindi deve essere particolarmente prudente. Le esperienze anche degli ultimi giorni le ricordo le strampalate dichiarazioni sui *social* del consigliere della Corte dei conti Marcello Degni, il quale si scaglia contro il Governo e critica l'opposizione perché non è stata sufficientemente energica nel contrasto al Governo in sede di legge di bilancio - richiedono, secondo me, degli interventi. C'è stato anche il caso della dottoressa Apostolico, che si era

sono pochi per definire un cronoprogramma. Posso rispondere subito che la prossima settimana il programma sarà illustrato alle Camere

due risposte. In primo luogo, per quanto riguarda le esternazioni dei magistrati, stiamo valutando anche degli interventi legislativi, perché hanno raggiunto livelli di intollerabile denigrazione dell'intero corpo della magistratura alcune esternazioni, sulle quali io ovviamente non mi pronuncio, ma si stanno già pronunciando gli organismi competenti. Credo che sia il minimo del buon senso ribadire il concetto quasi banale che i magistrati non solo devono essere imparziali, ma devono anche apparire tali. Se poi a questo aggiunge anche dei suggerimenti alla politica affinché intraprenda delle azioni che possano essere definite quasi eversive, beh, allora

ma c'è molto di più. Oggi noi siamo muniti di determinati strumenti: il cellulare non è più un documento, è una vita. Il suo cellulare non contiene solo le sue conversazioni con i suoi interlocutori, ma le conversazioni degli altri interlocutori con altri interlocutori, che vengono poi trasferite a lei attraverso quel sistema di inoltro (si chiama così) per il quale sequestrando un cellulare non dell'onorevole Zanettin (che non è sequestrabile) ma del signor Muzio Scevola, non si sequestra soltanto la vita di Muzio Scevola, ma anche quella di Furio Camillo, di Tizio, Caio, Sempronio e Martino. Noi stiamo sul *trojan* e anche molto oltre. È una situazione estremamente complessa, assolutamente nuova, che nei limiti del possibile sarà illustrata il 17 gennaio. I tempi di oggi sono quelli che sono,

Lo dico ancora una volta dopo averlo esposto l'anno scorso, anche se i giornali non ne hanno parlato perché le notizie che fanno notizia sono quelle brutte che sollevano polemiche. Noi stiamo intervenendo e siamo intervenuti, abbiamo avuto anche complimenti dei colleghi; abbiamo realizzato quello che era nei piani del PNRR, abbiamo ottenuto le rate, abbiamo rispettato i tempi e i metodi. Stiamo facendo di tutto per imprimere una velocizzazione, abbiamo ridotto l'arretrato. Il nostro cronoprogramma è di ridurre gli arretrati della giustizia civile, perché è l'incertezza del diritto, l'incertezza dei rapporti giuridici che incide economicamente sulla nostra vita finanziaria e poiché in questo momento l'emergenza maggiore è ancora purtroppo quella economica,

Signor Presidente, io mi dichiaro soddisfatto della risposta del Ministro, nella quale ho colto, sul piano dei contenuti, quei valori garantisti e liberali che lo contraddistinguono e che ci contraddistinguono in tanti anni di esperienza politica e di confronto che abbiamo avuto. Attendo pertanto con grande interesse quello che lei verrà a dirci la settimana prossima, raccomandandole a nome mio personale, dell'intera Forza Italia e credo di tutto il centrodestra, perché su questo siamo assolutamente uniti (in Commissione giustizia lavoriamo con grande sintonia con tutti i colleghi del centrodestra), quella grande svolta, quella grande riforma della giustizia che è tanto attesa. La riforma della giustizia, infatti, sembra una questione che riguarda solo gli addetti ai lavori, gli avvocati o i magistrati, invece è un tema sentitissimo, che l'opinione pubblica attende ed è un marchio di fabbrica, una connotazione specifica della nostra coalizione di centrodestra. Questa riforma l'attendiamo da tanti anni anche con riferimento alla memoria del nostro grande presidente Silvio Berlusconi e questa volta abbiamo l'occasione di farla. Credo che questo sia il momento giusto, il *timing* giusto: il Governo si è insediato da un anno, ormai ci conosciamo, collaboriamo insieme in maniera assolutamente sintonica e cordiale. La invito quindi a mettere il turbo ad arrivare presto nelle Commissioni giustizia di Camera e Senato, perché vedrà che i suoi provvedimenti saranno votati e apprezzati oltre che da noi, anche dai nostri elettori. *(Applausi)*.

elementare e militante antifascista, è rinchiusa in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza a Budapest, in attesa del processo con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti durante la manifestazione denominata Giorno dell'onore, un appuntamento durante il quale gruppi di estrema destra di tutta Europa si radunano in Ungheria. La Salis rischia una pena fino a sedici anni per lesioni gravi (anche se guarite in cinque e in otto giorni). Inoltre, le viene addebitato, senza alcuna apparente prova a suo carico, di essere legata a una organizzazione chiamata Hammerbande. Per lo stesso episodio, peraltro, e con gli stessi capi d'accusa, che, se confermati, nel nostro Paese porterebbero ad una pena massima di quattro anni, è attualmente agli arresti domiciliari in Italia Gabriele Marchesi, sul quale la Procura di Milano ha negato la richiesta di estradizione promossa dall'Ungheria, proprio in ragione della sproporzione della pena in relazione al fatto contestato. A Budapest, Ilaria Salis è sottoposta a condizioni di detenzione disumane: per sette mesi le è stato negato qualunque contatto con il mondo esterno, in un carcere nel quale, peraltro, i detenuti sarebbero legati sia ai polsi che ai piedi con cavigliere e in cui per il trasporto dei detenuti stessi verrebbe addirittura usato un guinzaglio di cuoio, per non parlare delle celle minuscole e sporche, della malnutrizione, dei gravi limiti all'igiene personale. Da tempo il padre di Ilaria Salis, che è stato proprio ieri qui al Senato per partecipare a una conferenza stampa organizzata dalla senatrice Cucchi, con diverse lettere ha sollecitato un intervento del Governo di fronte all'evidente violazione dei diritti umani che la figlia sta subendo: appello rimasto purtroppo senza esito. Signor Ministro, noi crediamo che il regime carcerario imposto dall'Ungheria sia del tutto incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti e le chiediamo se non ritenga assolutamente necessario doversi attivare immediatamente per promuovere l'applicazione delle convenzioni vigenti e avviare le procedure necessarie affinché la connazionale Ilaria Salis possa essere subito trasferita in Italia, trascorrere nel proprio Paese il periodo di custodia cautelare e partecipare al processo in videocollegamento, analogamente a quanto consentito al coimputato Gabriele Marchesi.

Il Governo italiano, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto di tutto per mitigare questa situazione. Alla prima udienza davanti all'autorità giudiziaria ha presenziato anche un funzionario dell'ambasciata, che si è interfacciato con il legale della ragazza. Il regime di detenzione è stato in parte limitato, nel senso che può adesso trattenere regolari colloqui con i familiari attraverso Skype. L'ultima visita consolare si è tenuta il 13 dicembre e sono state mitigate, nei limiti del possibile, le restrizioni di questa carcerazione severa. prevista la presenza di rappresentanti dell'ambasciata in qualità di osservatori alla prossima udienza del 29 gennaio. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, è inutile che ricordiamo che in assenza di una condanna definitiva, nessuna convenzione internazionale o un altro strumento consente l'esecuzione nel Paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario, quindi l'unico strumento vigente per noi è la risoluzione del 23 ottobre del 2009 del Consiglio giustizia e affari interni (GAI) sull'applicazione agli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e quindi non è applicabile nel caso concreto. Lasciatemi dire, purtroppo, che questo non è l'unico caso.

Noi ricordiamo - voi no, siete più giovani, ma io lo ricordo bene - il caso di Silvia Baraldini, che fu estradata dagli Stati Uniti con la solenne promessa che avrebbe scontato in Italia la pena che le era stata inflitta di oltre una volta arrivata in Italia, fu accolta con tutti gli onori all'aeroporto e poi scontò la pena in modo molto parziale. Gli americani questo lo ricordano ed è questo che ostacola, non solo con loro, le procedure che ogni volta noi cerchiamo di intrattenere, anche a livello fiduciario. Sotto questo profilo purtroppo, a causa di esperienze precedenti, la fiducia verso di noi è scemata. Questo non toglie - e concludo - che noi partecipiamo con grandissimo interesse e con grandissima attenzione attenzione al dolore dei familiari. Posso assicurare che faremo di tutto, nel rispetto delle regole e delle prerogative della giurisdizione nazionale e della giurisdizione internazionale, per mitigare la situazione di questa persona

*(Misto-AVS)*. Ministro, io ovviamente la ringrazio e capisco anche la complessità della vicenda. Però francamente non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto. Peraltro devo dirle che quello che è stato fatto dal Governo italiano mi sembra davvero molto al di sotto del minimo sindacale. Credo che, oltre a non essere soddisfatto io, non saranno soddisfatti proprio i familiari di Ilaria Salis, che per l'appunto chiedono al Governo italiano di intervenire su una vicenda che è davvero clamorosa dal punto di vista giuridico. Stiamo parlando di un carcere - lo ripeto - in cui non sono rispettati i diritti umani. Ieri Roberto Salis ha citato alcuni passaggi di una lettera drammatica della figlia, che scrive testualmente: «Sono rimasta cinque settimane senza ricevere il cambio lenzuola, sono stata costretta ad indossare abiti sporchi, malconci e puzzolenti, a indossare un paio di stivali con i tacchi a spillo, non ho potuto parlare con i miei avvocati e non ho potuto utilizzare un interprete». Io francamente, rispetto a questa situazione incredibile, che peraltro va avanti da undici mesi, quindi da un tempo significativo significativo e anzi molto ampio, penso davvero che non si possa semplicemente prendere atto di una questione complessa. Torno a chiederle, data la dimostrata e palese violazione dei diritti umani subita da Ilaria Salis, che il Governo si attivi proprio nel quadro della questione a cui lei ha fatto riferimento, cioè la decisione quadro 2009/829/GAI.

consentito all'altro indagato per i medesimi fatti (fortunatamente), perché la magistratura italiana stessa ha giustamente (io credo) rifiutato l'estradizione, proprio perché siamo dinanzi a una palese sproporzione. Parliamo purtroppo di una situazione in cui non sono rispettati i minimi diritti umani e io penso che il Governo debba fare tutto e anche oltre il possibile per salvaguardare i diritti umani di una propria concittadina che

una nuova finestra") *(M5S)*. Signor Ministro, la Commissione giustizia del Senato sta completando a passo di marcia, come se si trattasse di una priorità politica nazionale indifferibile, l'esame degli emendamenti al suo disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e il ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite. La quasi totalità degli esperti che sono stati auditi dalla Commissione giustizia ha evidenziato l'evanescenza delle motivazioni da lei addotte per questa riforma. La paura della firma non ha più alcuna ragion d'essere, tenuto conto che la riforma del reato di abuso d'ufficio del 2020 ha escluso radicalmente il sindacato del giudice penale su tutta l'amplissima gamma degli atti discrezionali della pubblica amministrazione. Quanto all'asserita inutilità del reato, che sarebbe dimostrata dall'elevato numero di archiviazioni e assoluzioni, le statistiche che sono state acquisite nel corso dell'audizione attestano che la percentuale media di archiviazione per tutti i reati è del 62 e che tale soglia è stata superata nel 2021 per le archiviazioni del reato di abuso d'ufficio, perché l'anno precedente, nel 2020, era stata approvata una riforma che ha depenalizzato tutta un'ampia gamma di comportamenti, che quindi sono stati archiviati. E un'ulteriore riprova dell'utilità del reato sono le 3.662 condanne definitive inflitte dal 1996 al 2020, una casistica impressionante di strumentalizzazioni affaristiche, nepotistiche e sopraffattrici delle funzioni pubbliche. Grazie alla sua riforma tutte queste condanne dovranno essere revocate. In sostanza, lo Stato e i cittadini onesti dovranno chiedere scusa a tutti questi abusatori conclamati per averli processati e condannati per comportamenti oggi ritenuti non più meritevoli di sanzione penale. A fronte del passo di marcia da lei impresso a questa e ad altre riforme, come quella in materia di intercettazioni, registriamo un'atarassica inerzia della maggioranza governativa a dare impulso ad altre riforme ripetutamente richieste dall'Unione europea e da altri organismi internazionali per colmare il divario tra l'Italia e e la quasi totalità dei Paesi europei in materia di regolazione delle *lobby*, di conflitto di interessi, strumenti essenziali di prevenzione della corruzione e per evitare che la politica si trasformi ogni giorno di più in cinghia di trasmissione di interessi di comitati di affari. È rimasto inascoltato il monito del Greco, l'organismo anticorruzione del Consiglio europeo, che ha rilevato che l'Italia, insieme all'Ungheria e alla Slovenia, è l'unico Paese europeo a non avere una legge sulle *lobby*. È rimasto completamente indifferente all'ultimo *report* dell'associazione Transparency, che ha denunciato che oggi sono 97 i deputati e i senatori portatori di interessi privati, che hanno cioè partecipazioni in aziende o ruoli in consigli di amministrazione. Tutto questo premesso, le chiedo, signor Ministro, se non ritenga opportuno togliere il piede dall'acceleratore delle riforme che aprono in vari modi ampi varchi al dilagare della corruzione e se, viceversa, non ritenga urgente accelerare l'intervento del Governo per addivenire, nel più breve tempo possibile, a un aggiornamento della legge in materia di conflitto di interesse, nonché a una legge che regolamenti l'attività delle *lobby*.

fatto (e ne faremo ancora), nelle nostre statistiche per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio. Ne parleremo più compiutamente un'altra volta, ma le assicuro che le cose non stanno come sono state da lei descritte.

Questo è vero, è un argomento serio e sarà trattato, perché - com'è noto - accanto alla riforma sull'abolizione del reato di abuso di ufficio, è già iniziata iniziata un'attività di concorso tra il Ministero e la Commissione presieduta dall'onorevole Buongiorno su una revisione, direi globale, dei reati contro la pubblica amministrazione, che è obsoleta, così come sono obsolete tante leggi. Ho fatto prima l'esempio del *trojan* e del cellulare, perché la tecnologia avanza in modo molto più veloce, così come avanzano in modo molto più veloce i sistemi della criminalità. Una volta mi sono permesso di dire che la mafia non parla per telefono; lei è stato molto severo su quello che ho detto, ma converrà che oggi la mafia dei sistemi, la vera mafia di comunicazione, noi non riusciamo nemmeno a intercettarla, perché sono così sofisticati che non abbiamo la possibilità di raggiungerli. È lì che dobbiamo concentrarci. Detto questo, per quanto riguarda invece le preoccupazioni dell'Europa sull'abuso d'ufficio, le posso assicurare che abbiamo studiato a fondo la questione. L'Europa non ci chiede l'introduzione o la reintroduzione del reato di abuso d'ufficio; ci chiede di combattere, secondo quanto ancora scritto nella Convenzione di Merida, la corruzione in tutte le sue manifestazioni. Sul punto noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è all'avanguardia, come lei sa perfettamente, dell'Europa sia per quanto riguarda le fattispecie sia per quanto riguarda la gravità delle pene. L'irrituale e l'improprio riferimento che si fa alla volontà dell'Europa fa invece riferimento a una proposta di direttiva che è in fase ancora molto embrionale e, quindi, è semplicemente una ipotesi su un'ipotesi che non sarà comunque trattata durante questa legislazione europea e che ha già sollevato parecchie critiche anche in altri Paesi, a cominciare dalla Germania.

comunque che il provvedimento sarà approvato quanto prima e posso assicurarle che non cederemo e non esiteremo di un pollice rispetto a quanto abbiamo fatto, detto e promesso.

comunicazione estremamente sofisticati; no, signor Ministro, noi abbiamo problemi con la mafia perché i mafiosi hanno capito che i soldi si fanno con i reati dei colletti bianchi, con il falso in bilancio, con l'evasione fiscale, con la corruzione. Hanno capito altresì che se non vogliono farsi processare e condannare, devono utilizzare gli stessi strumenti che i colletti bianchi hanno creato per garantire la propria impunità. Ormai c'è un termine corrente, si chiama mafia corruzione. Lei si ricorda il sacco edilizio di Palermo, quando hanno distrutto quella città? Quando in una sera concedevano 3.000 licenze edilizie? Lo sa come è stato fatto il sacco edilizio? Con l'abuso d'ufficio. Tutte queste licenze edilizie erano rilasciate infatti con l'abuso di ufficio. Proprio così. Il reato da contestare, oggi non lo potremmo contestare più. La mafia non fa più le estorsioni di una volta, ma si comporta come i colletti bianchi. Ha capito che bisogna farsi classe dirigente. Sono furbi. Perché rischiare con il traffico di stupefacenti e con le estorsioni non ricorrere a corruzione o concussione, grazie al fatto che la vostra maggioranza sta impedendo alla magistratura di portare alla luce questi reati con il *trojan*? Il *vulnus* alla *privacy*, il *vulnus* alla collettività al fatto che c'è una grande corsa alla distribuzione di 220 miliardi. Ci sono comitati d'affari, *lobby* e mafie che hanno il bavaglino, il coltello e la forchetta per la nuova corsa all'oro e in una fase come questa la maggioranza cosa fa? Da una parte dilata al massimo la discrezionalità incontrollata nell'affidamento di appalti pubblici multimilionari, abolisce il controllo concomitante della Corte dei conti, si prepara ad abolire quello successivo e lei cosa fa? Invece di rafforzare i presidi per evitare che questi soldi vadano a finire nel buco nero della corruzione e dello sperpero clientelare, normalizza l'abuso d'ufficio. Normalizza il conflitto di interesse. Lei normalizza il conflitto interesse perché abolisce l'abuso d'ufficio anche nella forma residuale che consiste nella violazione dell'obbligo di astenersi. Lei dice di no, ma è così. Noi diciamo al Paese, perché la politica criminale è una politica di orientamento culturale, che da questo momento in poi si può abusare del proprio potere, si può praticare il conflitto di interesse e poi ridimensiona, in una fase come questa, il traffico di influenze.

depenalizzando il traffico di influenze per tutte le utilità che non siano a carattere patrimoniale. Lei forse si sta occupando del problema della disoccupazione, perché aumenterà il numero dei lobbisti in modo assolutamente sproporzionato. Sotto questo profilo, il problema della disoccupazione di una parte significativa del malaffare l'abbiamo risolto.

quale sarà la percentuale che andrà agli affaristi, ai lobbisti, alla mafia? Non lo sapremo, ma certamente queste sue riforme contribuiranno ad alzare moltissimo questo livello percentuale.